Grazie,

Grazie,

L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un senatore Questore, che sarà effettuata a scrutinio segreto mediante schede. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, ciascun senatore potrà scrivere sulla propria scheda un solo nominativo.

Astore, Augello, Azzollini Baio, Balboni, Baldassarri,

Belisario, Benedetti Valentini,

Blazina, Bodega, Boldi,

Caligiuri, Camber, Cantoni,

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni,

Franco Paolo, Franco Vittoria Galioto,

Giordano, Giovanardi,

Lumia, Lusi Magistrelli, Malan,

Marinaro, Marini, Marino Ignazio,

Mazzaracchio, Mazzatorta, Mazzuconi, Menardi,

Sibilia, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speziali, Stancanelli,

Signor Presidente, colleghi, le voci critiche su questo provvedimento che l'Assemblea si accinge a valutare segnalano che mancherebbe un disegno organico e coerente di sostegno alla crescita economica e allo sviluppo produttivo del Paese. Noi siamo del parere che anche questo provvedimento, insieme agli altri che in questo triennio di legislatura sono stati adottati, si inscriva nella filosofia che ha governato la politica economica degli ultimi anni, che non poteva coltivare ambizioni di spesa a debito avendo il nostro Paese ereditato, come è noto, un debito pubblico che rappresenta il vero vincolo per uno sviluppo possibile. Dunque, si è scelta ancora una volta la strada della prudenza, della qualificazione dell'enorme spesa e della lotta all'enorme evasione, per recuperare risorse preziose per lo sviluppo. L'obiettivo del risanamento del bilancio pubblico non è una fissazione ragionieristica, ma è la condizione perché il Paese abbia la credibilità necessaria per agganciare lo sviluppo, che per la verità sta ripartendo nel mondo. Lo stesso obiettivo di equilibrio di bilancio per il 2014 non è illusorio, perché gli obiettivi di finanza pubblica di medio periodo, come hanno certificato tutti i maggiori istituti europei, si sono raggiunti, documentati dalla crescita dell'avanzo primario e dalla riduzione del deficit. Peraltro, il Piano italiano per la stabilità e per le riforme licenziato dal Parlamento nei mesi scorsi è stato valutato e apprezzato in sede europea. Nel corso della crisi l'Italia non ha attuato manovre di stimolo fiscale, che pur erano state da più parti sollecitate, non solo perché con il suo debito non poteva permetterselo ma anche perché sarebbe stato inutile fronteggiare una crisi globale con manovre anticicliche nazionali; sarebbe stata un traiettoria inutile e dannosa. Ci si è concentrati invece su misure che salvaguardassero la coesione sociale e il capitale umano del sistema produttivo, in attesa che la tempesta potesse passare. Anche i più critici ora sono portati ad osservare che quelle politiche hanno avuto successo. Il Paese non solo non ha messo ulteriormente a rischio i conti ma ha salvaguardato fattori decisivi, come la pace sociale e il capitale umano delle imprese, che poi rappresentano l'aspetto portante del sistema produttivo italiano. Certo, restano sullo sfondo i temi della crescita debole e dei fattori strutturali che da anni rallentano le dinamiche espansive della nostra economia. Le manovre di questi anni non potevano influenzare le debolezze strutturali del nostro sistema, con la conseguenza di bassi tassi di occupazione, soprattutto tra i giovani, le donne e nel Mezzogiorno. Questo è il compito che oggi va ripreso con realismo, ma anche con audacia. Siamo consapevoli, colleghi, che questi obiettivi, crescita e lotta alle disuguaglianze, rappresentano la cifra e il senso di questa seconda parte di legislatura. il contesto europeo anche in questo provvedimento resta il riferimento ineludibile. Infatti, il decreto‑legge si ricollega non solo nel suo titolo alle procedure previste nell'ambito del cosiddetto semestre europeo, in base al quale la sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali si articola in una serie di fasi che prevedono la presentazione contestuale da parte degli Stati membri dei programmi di stabilità o di convergenza e dei programmi nazionali di riforma. Siamo quindi inseriti in una logica di coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche, per cui gli Stati membri si impegnano ad adottare misure necessarie per stimolare la competitività e l'occupazione. Tutto ciò si ricollega alla Strategia di Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, definita dal Consiglio europeo nel giugno 2010, che inserisce tra gli obiettivi principali il miglioramento delle condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare l'obiettivo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati nel settore della ricerca. Il decreto si muove nella linea, costantemente affermata dal Governo, della priorità da assegnare ai vincoli di bilancio, linea ancora recentemente confermata nel Documento di economia e finanza. Il rispetto dei saldi è obiettivo ineludibile, come abbiamo detto, e si rivela tanto più essenziale oggi, in una fase nella quale, a seguito delle turbolenze in materia di finanza pubblica emerse in alcuni Paesi dell'eurozona in attuazione del Patto euro plus, sarà necessario per l'Italia porsi l'obiettivo di una progressiva riduzione del rapporto tra debito e PIL, da perseguire attraverso il permanere del controllo sui saldi e insieme attraverso politiche che accentuino i ritmi di crescita del prodotto interno. Non sfugge dunque a nessuno che questo è solo il primo di una serie di decreti che rientrano in quella logica europea del semestre. Proprio quegli impegni ci obbligano a perseguire l'obiettivo più difficile: attuare le riforme per il rilancio della competitività senza gravare il bilancio pubblico: un cammino certo difficile per un traguardo che non è raggiungibile con un editto. Per questo il provvedimento fa perno su tagli degli adempimenti burocratici, sulla semplificazione, sullo snellimento di procedure, sulla riduzione di obblighi amministrativi, sull'abolizione della duplicazione di controlli: tutte misure senza oneri a carico dello Stato. Gli interventi in ambito fiscale sono di sicura rilevanza: tra i più importanti ricordiamo il credito d'imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno Mezzogiorno e quello per gli investimenti nella ricerca, per tentare di raggiungere l'obiettivo di cui abbiamo parlato; la riduzione degli obblighi di comunicazione e razionalizzazione dei dei pagamenti; la regolamentazione delle verifiche degli accessi; le semplificazioni per i contribuenti con contabilità semplificata e così via, passando per l'accelerazione delle opere pubbliche e per il rilancio dell'edilizia privata; l'assunzione dei precari nella scuola; l'ampliamento dei servizi telematici ai cittadini; il rilancio della nautica da diporto; il potenziamento dei distretti turistici; la prosecuzione del progetto della Banca del Mezzogiorno, con l'autorizzazione all'emissione di titoli di risparmio per 3 miliardi di euro con facilitazioni fiscali per i sottoscrittori. Certo, c'è ancora molto da fare. C'è da dare una risposta alle famiglie, e vi è l'enorme tema della riforma fiscale nel suo complesso, ma non vi è di certo argomento per essere radicalmente contrari, né pessimisti su questo provvedimento. L'opposizione, nel corso del dibattito, franco è svolto in Commissione in questi giorni, ha spronato il Governo e la maggioranza su alcuni problemi che a nostro modo di vedere meritano sicura considerazione, pur di fronte alla complessità delle soluzioni: il tema dello smaltimento dei debiti della pubblica amministrazione, attraverso un veicolo societario costituito dalla Cassa depositi e prestiti;

sulle procedure per l'appalto delle opere pubbliche che, pur dovendo conseguire obiettivi di velocizzazione, non possono abdicare alla necessaria esigenza di trasparenza e di concorrenza.

tentativi di semplificazione, specificando che si tratta comunque di azioni che si inseriscono in un processo già avviato da tempo e che deve proseguire per sostenere la competitività del nostro sistema industriale.

misure che sostengono peraltro il nostro sistema pubblico di ricerca e le sue importanti competenze dislocate in diversi poli sul nostro territorio nazionale. C'è ancora certamente molto da fare per quanto riguarda il tema del Mezzogiorno: in particolare, ritengo che i provvedimenti efficaci per lo sviluppo del Sud debbano riguardare la fiscalità di vantaggio, a beneficio di un rilancio degli investimenti e della produttività, la vera «palla al piede» della nostra economia. Per questo, le misure dell'articolo 2, riproponendo il credito d'imposta per un nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, potranno dare un contributo rilevante e segnare anche una traccia che deve incoraggiare il negoziato, sia con l'Unione europea che con le Regioni, per un impiego più efficace delle stesse risorse europee.

deve essere affrontata dal Governo nonché da tutte le componenti politiche e istituzionali del nostro Paese con la massima attenzione e con una grande consapevolezza. A ciò provvede in via definitiva la manovra che sarà a breve all'esame di quest'Aula. Si tratta di un passaggio cruciale, che condizionerà le prospettive economiche e politiche della stessa Unione e inciderà sulle opzioni di politica economica di lungo periodo per gli Stati membri.

Signor Presidente, con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il Governo ha realizzato una serie di misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia, allo scopo di riavviare lo sviluppo del sistema Paese senza appesantire i conti pubblici avviati verso

del provvedimento e la volontà del Governo rispetto ad un intervento importante come quello dello sviluppo. Beneficeranno di questo decreto numerose categorie: dalle grandi alle piccole e medie imprese, dalle famiglie ai liberi professionisti,

le famiglie italiane. Sarà possibile riconvertire il mutuo di casa da tasso variabile a tasso fisso; il mutuatario potrà rinegoziare il proprio mutuo; il tetto del mutuo rinegoziabile è di 150.000 euro. Novità importanti

identità. Semplificazioni si riferiscono anche alla comunicazione dell'aggiornamento dei carichi di famiglia: non sarà più obbligatorio comunicare al sostituto d'imposta l'aggiornamento se non ci saranno variazioni. quanto riguarda le piccole e medie imprese, arriva l'estensione della contabilità semplificata: la misura coinvolgerà le imprese di servizio e altre imprese. Si procederà a semplificazioni di tipo amministrativo e sgravi fiscali anche per i distretti turistico-alberghieri.

del Meridione. Dal 2011 al 2013, l'imprenditore che vorrà assumere un lavoratore tempo indeterminato potrà beneficiare di un credito d'imposta pari a 300.000 euro per ogni lavoratore assunto. Novità si registrano anche per i controlli amministrativi sulle aziende, che potranno essere, da ora in poi, solo a cadenza semestrale e potranno durare al massimo 15 giorni: la violazione di tale misura costituirà un illecito a livello disciplinare. Nuove misure si registrano anche nell'ambito della ricerca per le aziende italiane. Anche il Ministero dalla pubblica istruzione, e non solo quello dello sviluppo, sarà autorizzato a stipulare contratti con soggetti privati e pubblici per programmi di ricerca.

In questo beneficio sono comprese categorie importanti come gli atenei statali, gli istituti universitari legalmente riconosciuti (statali e non statali), gli enti pubblici di ricerca, l'ASI (l'Agenzia spaziale italiana) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. All'articolo 2 si prevede la concessione di un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto stabilmente nel Mezzogiorno (nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia). Ciò al fine di incrementare il livello occupazionale nel Mezzogiorno attraverso l'erogazione di un incentivo fiscale concesso nella forma del credito d'imposta. Nella sostanza, la disposizione tende a ridurre il costo del personale, stimolando il mercato del lavoro: Il credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi salariali, sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, se il lavoratore è svantaggiato.

All'articolo 2-*bis* è previsto il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, finanziato con Fondi strutturali europei. All'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere istituiti nei territori costieri, su richiesta delle imprese turistiche che operano in quei territori,

In base alle modifiche apportate dalla Camera, la delimitazione dei distretti turistici non è più effettuata dall'Agenzia del demanio ma dalle Regioni, d'intesa con i Comuni interessati. Quindi, il territorio viene coinvolto in maniera diretta attraverso la conferenza dei servizi, a cui deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Sempre in quest'articolo, al comma 7, si affronta il tema della semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali, senza

L'articolo 4 merita una trattazione e un approfondimento a parte perché contiene una serie di semplificazioni per la realizzazione delle opere pubbliche, garantendo l'efficacia dei sistemi di controllo. Nel campo delle costruzioni, in particolare, viene effettuato un doppio intervento di semplificazione indirizzato, da una parte, allo snellimento delle procedure di autorizzazione in materia di edilizia privato e, dall'altra, alla riduzione dei tempi di

i lavori con la procedura negoziata senza bando di gara a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,

semplifica i procedimenti di appalto delle opere minori, ma garantisce anche il lavoro alle piccole e medie imprese che, altrimenti, verrebbero sopraffatte da quelle grandi. Lo spirito di questa disposizione è: spendere meglio e più rapidamente. di un decreto-legge che senz'altro interviene trasversalmente su molte materie, ma incide profondamente soprattutto nella materia delle opere pubbliche, apportando una serie di modifiche al codice dei contratti pubblici, peraltro recentemente esaminato e modificato dall'8a Commissione. Si tratta, tuttavia, di modifiche che il Governo ha ritenuto indispensabili e improcrastinabili ai fini della riforma amministrativa, volta alla semplificazione dei procedimenti, alla riduzione delle lungaggini burocratiche attualmente esistenti e, soprattutto, alla riduzione dei costi sia per gli operatori economici che per la pubblica amministrazione. Passando ad esaminare l'articolo 5, esso introduce modifiche importanti alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata, sempre con la finalità di apportare snellimenti procedurali. Si segnala in questo articolo un altro aspetto rilevante, consistente nel ricorso ad una maggiore informatizzazione dello Sportello unico per l'edilizia. unico per l'edilizia. Tra le principali modifiche apportate dalla Camera si prevede, inoltre, la soppressione delle disposizioni riguardanti l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, purché funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, a carico del titolare del permesso di costruire. Si tratta di una grave perdita di una norma importante di semplificazione dovuta all'approvazione

ai commi 1 e 2, per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese il decreto ha apportato alcune importanti modifiche, che mi permetto di elencare, in quanto servono a caratterizzare il provvedimento: le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e quindi non trovano applicazione nei rapporti tra le imprese; la pubblica amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e dei documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; privato; la riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL; la facoltà di effettuare *on line* qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini; per i trasporti eccezionali, l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata. L'articolo 7 reca un complesso di norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in diversi ambiti. L'articolo 8, al comma 1, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003, e specificamente alla tipologia del contratto d'inserimento, al fine di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro delle donne prive di un regolare impiego da almeno sei mesi.

ritardati pagamenti dei debitori dalle banche dati sui rischi creditizi, ovvero a cancellare le segnalazioni se il debito non è superiore a sei rate mensili o a un'unica rata semestrale.

dello sviluppo economico, a stipulare appositi accordi di programma per la ricerca strategica con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, e con distretti per realizzare interventi di programmazione negoziata volti a valorizzare prevalentemente le aree sottoutilizzate e il Sud.

unificazione della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato.

quello contenuto nel decreto-legge all'articolo 4, di cui poi parlerò, e ad inserire una nuova misura che riguarda i crediti delle imprese con la pubblica amministrazione.

Da parte della maggioranza e del Governo però è venuta una risposta negativa. Credo allora che innanzitutto, prima di esplicitare le proposte del Partito Democratico su questo provvedimento, dobbiamo porci la domanda del perché abbiamo avanzato questa iniziativa politica. Ebbene, l'abbiamo proposta per dare un senso a questo provvedimento

di tutta la stagione della manovra che stiamo cominciando in questi giorni a vedere, per ora soltanto dalle indiscrezioni giornalistiche. Quindi, c'è un *link* preciso tra il decreto sviluppo e la manovra che nei prossimi giorni arriverà all'esame del Senato. Infatti, l'Italia - non la maggioranza, o il Governo - si muove in uno stretto percorso:

intanto delle forze produttive italiane, e soprattutto necessiterebbe di un percorso chiaro da parte del Governo e della maggioranza. Il cosiddetto decreto sviluppo avrebbe dovuto cominciare a declinare i termini delle misure che sostengono la crescita italiana: favorire la competitività delle imprese, dare uno stimolo effettivo alla produttività dell'economia italiana, intervenire dunque sull'economia reale. Per chi lo avesse dimenticato, questo era il decreto che avrebbe dato la scossa all'economia italiana; non so se ricordate la conferenza stampa in cui il presidente Berlusconi parlò di questo provvedimento come quello che avrebbe dato la scossa all'economia italiana. italiana. Su cosa incide effettivamente il decreto? Il risultato, a dire il vero, è perfino imbarazzante. Il provvedimento è sostanzialmente vuoto, se si eccettua il credito d'imposta per la ricerca, su cui mi soffermerò tra breve. Il provvedimento ripropone in maniera del tutto appassita ed inefficace la filosofia alla base delle vecchie scelte di politica economica del centrodestra italiano, cioè un *mix* di alleggerimento delle regole. Qui di regole se ne alleggeriscono molte, in primo luogo in materia di appalti, in materia fiscale, in materia urbanistica e nelle modalità della riscossione coattiva. Tutto ciò non ha niente a che vedere - mi rivolgo ai colleghi relatori di maggioranza - con la semplificazione e la velocizzazione dei provvedimenti: va in una direzione esattamente opposta, e in alcuni casi rischia di generare persino danni. Questa miscela è è quella che ha fatto fallimento negli ultimi tre anni di governo del centrodestra, perché altra è la natura dei problemi che l'Italia ha di fronte. Entrando nel merito,

Non mi soffermo su alcuni aspetti che sono anche positivi e vanno effettivamente nella direzione di un alleggerimento e di un'accelerazione delle procedure, ma mi soffermo piuttosto su un aspetto particolarmente preoccupante. Mi riferisco, in particolare, Mi riferisco, in particolare, ai commi e alle lettere dell'articolo 4 che riguardano l'affidamento senza gara dei contratti di lavoro cosiddetti sotto soglia comunitaria

Credo che questo sia un fatto straordinariamente grave, perché la conseguenza è duplice. La prima è sul versante dell'etica pubblica e della trasparenza. Mi permetto di dire - e lo dico in maniera un po' brutale - che rischiamo in questo modo di fare una sorta di nazionalizzazione della cricca, cioè di stabilire un principio in base al quale si va ad una opacizzazione totale delle procedure di appalto. La seconda conseguenza forse è persino più grave, perché è di carattere economico. Le imprese italiane vengono spinte non alla competizione tra di loro, ma al capitalismo relazionale di carattere locale serve a dire alle imprese che è più importante andare a cena al circolo del golf con il sindaco, con il direttore delle associazioni imprenditoriali, piuttosto che stare sul mercato a combattere, con la conseguenza che quando quelle imprese si sposteranno di qualche chilometro dal luogo della loro residenza saranno completamente fuori mercato. L'Italia purtroppo è piena di questi esempi. Aggiungo che la valutazione che voi fate che questo provvedimento servirebbe a dare maggiore velocità viene smentita dai fatti. Nel 2008 questo Governo e questa maggioranza hanno alzato la soglia senza gara dai 100.000 euro ai 500.000 euro. Basta guardare i fatti ed è evidente che dal 2008 non solo non c'è stata alcuna accelerazione nei tempi di realizzazione delle opere, ma addirittura, anche a seguito della clamorosa caduta degli investimenti e della spesa in conto capitale, le opere italiane sono nella condizione che tutti conoscono. Così non va, Così non va, perché tutto questo è un fatto grave che - come dicevo - va a colpire direttamente la concorrenza e la competitività delle imprese italiane. L'esatto opposto di quello di cui ci sarebbe bisogno e che viene detto anche nei documenti del Governo. Il secondo punto - poi vado rapidamente ad altre considerazioni - riguarda il sistema della riscossione, che viene anch'esso profondamente modificato: sto parlando della riscossione coattiva. al riguardo, non c'è dubbio che ci fosse bisogno - ed è stato detto correttamente dai colleghi relatori - di rideterminare le modalità della riscossione coattiva da parte di Equitalia. Abbiamo portato molti esempi, anche nel dibattito di Commissione, sulla sproporzione tra l'ammontare della riscossione e le esecuzioni che Equitalia mette in campo: non c'è dubbio che bisogna fare questo, ma da qui a quello che prevede il provvedimento ce ne passa. Per essere obiettivo, vorrei leggere qualche passaggio di una lettera che è stata inviata ai colleghi senatori dal presidente e dal vice presidente dell'ANCI (quindi non faccio una valutazione di parte). In questa lettera si dice che le misure che sono contenute nel provvedimento del Governo sono pericolose per la sicurezza delle entrate comunali e incoerenti rispetto al processo di attuazione del federalismo attualmente in corso pericolose per la sicurezza delle entrate comunali). Questo, oggi, quando tra l'altro il Governo, come sappiamo, con la manovra colpirà ancora in maniera forte esattamente le disponibilità degli enti locali perché - aggiungono i firmatari di questa lettera - la maggior parte delle posizioni della riscossione si attesta su importi inferiori ai 2.000 euro. Allora, si aggiunge, è utile il ripensamento del ruolo svolto da Equitalia, ma questi provvedimenti rischiano di generare una frammentazione clamorosa della riscossione, e soprattutto fanno uscire Equitalia dalla riscossione di questi importi, spingendo alla creazione di nuove società pubbliche *in house* presso gli enti locali. Pensate che splendida conclusione, e che semplificazione! Abbiamo detto tutti che uno dei punti da aggredire anche nella prossima manovra - noi lo faremo come Gruppo del Partito Democratico - sono le oltre 7.000 società pubbliche di carattere locale, che non danno certo un contributo alla semplificazione e alla produttività, e in questo modo si va nella direzione opposta, sollecitando, spingendo e persino obbligando gli enti locali a costituire delle nuove società pubbliche nel settore della riscossione, mettendo tra l'altro gli enti locali di taglia più piccola in una condizione naturalmente drammatica: infatti, mentre alcuni enti locali avranno le capacità tecniche e le risorse anche professionali, oltre che economiche, per andare incontro a questo problema, gli altri, la stragrande maggioranza degli enti locali, con qualche considerazione aggiuntiva. Noi, con i nostri emendamenti, che hanno un profilo molto chiaro e preciso e che danno l'evidenza di una linea politica e di politica economica in questa materia,

per le erogazioni che vengono fatte alle università - sostanzialmente di questo si parla - ma si dovrebbe incardinare meglio sulla vicenda industriale dell'impresa il tema della ricerca. Un esempio per tutti: un prototipo rientra in questo discorso? seconda considerazione riguarda la stabilizzazione dei crediti d'imposta del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici come dato strutturale di fondo. affrontata dai nostri emendamenti è la riduzione dell'IRAP, eliminando il costo del lavoro dalla base imponibile. Il quarto punto riguarda interventi a sostegno delle infrastrutture.

L'Italia non ha bisogno di questi colpi di teatro. L'Italia non ha bisogno di annunci e di grandi improvvise svolte che non si realizzeranno mai, perché l'economia di oggi non funziona così: per questo le ricette del centrodestra non fanno non fanno ripartire minimamente la crescita del Paese. C'è bisogno, invece, di un lavoro paziente, tenace. Non ci sono scosse da dare. Bisogna fare uno sforzo di sistema, richiamare tutte le energie del Paese, e sono tante, ad uno sforzo solidale. Faccio anche in questo caso un esempio: non ci si deve preoccupare di far entrare qualcuno nel sistema riservato degli appalti, a fronte di ogni imprenditore che entra in quel sistema ce ne sono 10, 100, 1.000 che al mattino tirano su la saracinesca, si rimboccano le maniche e lavorano e cercano di stare sul mercato. Noi del Partito Democratico vogliamo guardare a quegli artigiani, a quei commercianti, a quei piccoli imprenditori che tutti i giorni fanno i conti con i problemi dell'economia e della competizione. Questo è un provvedimento macchinoso, confuso, in qualche caso anche pericoloso. Soprattutto, è un provvedimento improduttivo di positivi effetti concreti. D'altronde, signor Presidente, non è servito nemmeno a farvi prendere qualche voto alle elezioni.

perché, ripeto, non funziona. Non credo quindi che sia il caso che questo ramo del Parlamento si limiti ad un esame burocratico,

sul provvedimento, ma lo farete non certo per l'atteggiamento dell'opposizione. I nostri emendamenti, come è stato riconosciuto anche dai colleghi relatori di maggioranza, sono tutti molto di merito, molto precisi e privi di qualsiasi carattere ostruzionistico. Metterete la fiducia semplicemente perché avete paura di affrontare le questioni che noi abbiamo posto.

Restano confermati gli argomenti già presenti in calendario per la settimana corrente. La settimana dall'11 al 15 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, con particolare riferimento al decreto-legge in materia di stabilizzazione finanziaria. Al fine di consentire congrui tempi di esame alla Camera dei deputati, la discussione in Assemblea del predetto provvedimento inizierà nella seduta pomeridiana di martedì 19 luglio, alle ore 17, per concludersi entro la giornata di giovedì 21. Per garantire il più ampio dibattito, la durata delle sedute è stata ampliata rispetto ai consueti orari. Il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione bilancio. è in corso la votazione a urne aperte per l'elezione del senatore Questore. Le urne resteranno aperte sino alle ore 12,30; successivamente si provvederà allo scrutinio e alla proclamazione del senatore Questore eletto. **Programma

L'ordine del giorno reca la votazione sulle dimissioni ripresentate dal senatore Nicola Rossi con lettera del 9 febbraio 2011 a seguito del voto dell'Assemblea in data 2 febbraio. Do lettura dell'ultima lettera inviata dal senatore Rossi il 30 giugno scorso: «Caro Presidente, nella prossima settimana l'Aula si esprimerà circa la richiesta di dimissioni di cui alla mia del 9 febbraio, u.s. Per evidenti motivi di opportunità non sarò presente alla seduta. Le sarò grato, peraltro, se vorrà informare l'Aula del fatto che la mia assenza sarà da intendersi solo ed esclusivamente

il via, signor Presidente.

Grazie, signor Presidente. Vorrei solo chiedere ai colleghi un momento di riflessione sulla decisione che dovremo assumere come Indubbiamente, nella sua coerenza il collega Nicola Rossi ha mantenuto la sua volontà di rassegnare le dimissioni da quest'Aula. Io credo però che l'Aula debba respingere queste dimissioni,

Forse in questo momento, in cui noi tutti, come classe politica, siamo soggetti, da parte dell'opinione pubblica, a giusti, o meno giusti, rilievi critici,

che certamente hanno un fondamento solido di verità - e cioè di riconoscimento del valore della qualità dell'impegno politico e civile

per dare luogo a questo suo gesto. E se se ne accettano le motivazioni, francamente diventa difficile difendere al di fuori di quest'Aula il ruolo dello stesso Senato. Se si respingono le dimissioni del collega Rossi, si respingono anche le sue motivazioni, cioè si dà un segno di speranza a questo Paese nel si può continuare a combattere per le proprie idee in trasparenza nell'Aula più alta di rappresentanza istituzionale della Repubblica italiana. Per questo, cari colleghi, vi chiedo un attimo di riflessione,

Presidente, la mia purtroppo ormai lunga esperienza di Senato mi ha indotto a concludere che ci sono due tipi di lettere di dimissioni. Ci sono coloro che si sono dimessi e hanno mandato una lettera affinché questa venga accettata e ci sono coloro che si sono dimessi e hanno mandato una lettera affinché questa sia respinta (questa mia esperienza copre anche casi di richieste di dimissioni reiterate).

apre una nuova finestra"). Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Nicola Rossi.

tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

come ha ben evidenziato già il senatore Agostini, ed è anche desumibile da molte valutazioni espresse nel dibattito in Commissione dagli stessi relatori di maggioranza, risalta con tutta evidenza il problema della totale incertezza relativamente ai profili e agli effetti finanziari che potranno derivare dalle singole disposizioni contenute nel decreto-legge in esame e, più sinteticamente, dal provvedimento nel suo complesso. elemento dell'ormai lunga sequenza di provvedimenti *omnibus*, che ha sì un titolo pretenzioso, «Prime disposizioni urgenti per l'economia», evocando appunto il collegamento con la manovra che verrà e che discuteremo dalla prossima settimana in quest'Aula del Parlamento, ma che poi si disarticola in una varietà di materie e ambiti tra loro poco raccordati e disomogenei. Io non nego che siano da considerare come apprezzabili le disposizioni sul credito d'imposta per sostenere la ricerca scientifica e la collaborazione imprese-università, come pure le disposizioni sul credito d'imposta a sostegno delle nuove assunzioni nel Mezzogiorno per i giovani: sono misure che già aveva varato nella XV legislatura l'allora Governo Prodi, ed è una grave, colpevole responsabilità questo segnale di tardiva resipiscenza da parte della maggioranza. la traduzione operativa di queste intenzioni è suscettibile di generare disparità di trattamenti e non certo a favore di chi maggiormente ne potrebbe vantare merito (penso alle imprese che hanno investito nei due anni precedenti al 2011, quelli in cui era più arduo e complicato farlo) e anche il richiamo ai*placet* dell'Europa perché le misure sull'occupazione nel Mezzogiorno possano diventare operative suona molto come un'astuzia dilatoria.

gli incentivi previsti sono puramente organizzativi, di portata finanziaria modesta, e con i limiti e le contraddizioni che ho evidenziato. Ma se le luci di questo sedicente decreto per lo sviluppo sono fioche, le ombre sono invece corpose: penso a tutte le discutibili innovazioni con cui riformate la normativa sugli appalti, su cui si è già soffermato ampiamente il relatore di minoranza, stigmatizzando sia i rischi di opacità nelle procedure individuate per lo svolgimento delle gare pubbliche sia il pericolo di abbassare ulteriormente il livello e la capacità competitiva, a scapito delle imprese più dinamiche e capaci. Anche le misure sulla semplificazione fiscale e burocratica, che pure sarebbero pienamente condivisibili, si connotano per profili che favoriscono più le convenienze di soggetti economici forti (penso alle banche e alle imprese di costruzione), a spese della tutela del territorio, di qualche corposo aspetto di equità e legalità, dell'interesse dei consumatori. Mi soffermerò più analiticamente riguardo alle disposizioni in materia di semplificazione fiscale, perché esse costituiscono in qualche modo una spia rivelatrice di un'impostazione che ritroviamo, purtroppo, in tutta la politica economica seguita dal ministro Tremonti. Certo, ben venga la semplificazione, ci mancherebbe altro. Nel decreto si dispone l'unificazione del controllo amministrativo e si impongono tempi più stringenti a chi deve operare: le autorità pubbliche non potranno effettuare più di un controllo a semestre; potranno guardare i conti, certo, ma non tenere l'azienda sotto osservazione per più di 15 giorni. Ma è proprio qui che cominciano i dubbi per come è costruita la norma. Si arriva al suggerimento davvero un po' singolare e strano, di cui non so se ve ne era davvero bisogno (non è mortificante e offensivo secondo il quale gli operatori della Guardia di finanza, quando possono, si debbono presentare in borghese a svolgere i loro compiti. Le norme sono costruite in modo che le disposizioni sui controlli e gli accessi degli operatori fiscali sembrano più rispondere all'esigenza di un manifesto di propaganda politica per intercettare e surrogare a buon mercato un disagio che tanti artigiani e piccoli imprenditori soffrono per le difficoltà della situazione economica, segnalando l'amministrazione finanziaria come fosse un «altro da sé» rispetto al Ministero competente e al Governo, e dunque un responsabile su cui scaricare e censurare i comportamenti, con un'intenzione più deteriore sottesa a questa prima presa di distanza e cioè mandare un segnale e determinare di fatto un ambiente e un clima per chi deve operare in cui sia più forte la propensione ad alleggerire gli accertamenti e le ispezioni. E qui rispunta il nervo scoperto di questa maggioranza e delle politiche fiscali del ministro Tremonti. Il contrasto all'evasione fiscale richiede una linea di rigore e di coerenza, rispetto e tutela dei diritti del contribuente, correzione di distorsioni quando e per i casi in cui l'agire dell'Agenzia o di Equitalia è troppo invasivo, sproporzionato e vessatorio; ma non ci può essere nessuna incertezza sulla pretesa dell'ottemperanza da parte di ciascun soggetto contribuente, alle proprie obbligazioni fiscali. È così che si costruisce un atteggiamento e una propensione al rispetto della legalità e del rapporto corretto di lealtà dei contribuenti nei confronti del fisco. Il modo in cui, invece, è trattata la questione della riscossione in questo provvedimento contraddice e svalorizza questi principi. Va detto che, nella logica che ho ricordato, la riscossione è chiamata ad assolvere a un ruolo forse ingrato, ma sicuramente importante e necessario.

La quantità di tributi riscossi è raddoppiata in questi anni: forse avrà urticato qualche contribuente recalcitrante, ma il risultato è da apprezzare, anche perché siamo ancora molto al di sotto della elevata quantità di ruoli che risultano nei residui attivi dello Stato e di molti enti pubblici, che devono quindi essere recuperati. Probabilmente andrebbero sottoposti a valutazione per quota parte anche quelli che sono in una condizione di effettiva consistenza ed esigibilità, ma proprio per questo il lavoro di Equitalia è da incoraggiare, non da limitare o da ostacolare. Il che naturalmente non significa che non ci siano miglioramenti da adottare, procedure da rivisitare, soglie che fanno scattare ingiunzioni e pignoramenti da riparametrare per salvaguardare le finalità e e mantenere la correttezza delle relazioni tra contribuenti e fisco. Ma questo è il compito del legislatore e gli emendamenti che noi abbiamo presentato in proposito avevano proprio questa ispirazione e penso che, se fossero stati accolti, avrebbero aiutato a conseguire il risultato che ho richiamato. Sul tema della riscossione, però, anche per effetto delle altre norme adottate in materia con questo provvedimento, bisognerà ritornare con un approccio più sistemico e una visione più equilibrata ed organica, perché la scelta di "scaricare" Equitalia di una forse fastidiosa incombenza e di riportarla in capo ai Comuni, che dovranno organizzarla già a partire dal 1° gennaio 2012, è foriera di conseguenze che non saranno indolori. Innanzitutto, alcuni riflessi graveranno già sul bilancio 2011 di molti enti locali, che potevano aver stimato (come penso abbiano fatto), in forza del *trend* consolidatosi, una previsione di entrate da riscossione coattiva che non si realizzerà; luogo, molti Comuni si troveranno impreparati e con armi anche più spuntate nell'esigere il rispetto delle sanzioni comminate, con pregiudizio al solito del civismo e di chi adempie correttamente alle proprie obbligazioni tributarie. Naturalmente non ci sfugge che anche in questo ambito possano essersi determinate grossolanità nei comportamenti di Equitalia, atteggiamenti da correggere e situazioni da registrare, attraverso una migliore «presa in carico del problema», in un rapporto di miglior coordinamento con le amministrazioni di riferimento, che hanno certo strumenti e sensibilità per ammortizzare le situazioni meritevoli di aiuto e graduazione, ma non possono essere lasciate a se stesse quando si tratta di sanzionare ed esigere il rispetto della legalità e del civismo.

questo lasciar spazio al «fai da te» avrà l'effetto di far proliferare società *in house* o rapporti di affidamento in concessione che aumenteranno i costi passivi e non è detto che incrementino l'efficacia. Né vale trincerarsi dietro il paravento di un'autonomia lasciata ai territori, in nome di un federalismo che perde i pezzi e subisce colpi ad ogni passaggio parlamentare, perché si sarebbe potuta collocare una riflessione complessiva sul tema della riscossione, prevedendone la messa a regime nel momento della sua entrata in vigore, dal 2014, approfittando così di questa fase transitoria per una più meditata e partecipata messa a punto. Infine, si apre un serio problema anche dal punto di vista delle ricadute complessive sui saldi di bilancio, di cui pare nessuno, né al Governo, né nella maggioranza si preoccupi. Ma di questo non vi occupate, perché ci sarà sempre un ente locale o qualche categoria di imprese e contribuenti reali su cui far gravare gli effetti della vostra disinvoltura, dei vostri pasticci, dei vostri errori. Lo avete già fatto anche con questo provvedimento: vedi l'introduzione della possibilità di revisione retroattiva delle classificazioni catastali ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili e della conseguente esclusione dall'ICI, tema assai disputato e controverso, rispetto alla quale non c'è da parte nostra contrarietà ed anzi spesso lo avevamo auspicato e sostenuto. Ma il punto è che non si possono scippare in corso d'anno risorse già iscritte in entrata da parte dei Comuni, senza avvertire l'esigenza di una valutazione e compensazione. È comodo farsi belli con la faccia degli altri, e soprattutto è inaccettabile mettere altri, come avete fatto con il provvedimento sul federalismo municipale, nella condizione di assumere misure impopolari per conto terzi. In questi anni quel Robin Hood che aveva iniziato la legislatura si è perso nella foresta e ha lasciato campo vinto al principe Giovanni e alle sue prepotenze e crudeltà. Il problema per voi adesso è però che finalmente un bel po' di opinione pubblica se n'è accorta, e non vi riesce più di approntare camuffamenti e di fare ricorso a quella spregiudicata operazione di distrazione di massa a cui ci avete abituato. Certo, oggi porrete la fiducia e approverete questo provvedimento, comprimendo per l'ennesima volta lo spazio di un confronto parlamentare. Si butta via un'occasione. Vi avevamo sollecitato a concentrare su alcuni punti qualificanti la discussione, e in particolare sul tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese creditrici. Sarebbe bastato almeno questo, anche parzialmente inserito, a dare un senso, una finalità, un'anima a questo decreto-legge. Ci dobbiamo rassegnare a un pur importante ordine del giorno, ottenuto in Commissione, che impegna il Governo a inserire nella manovra che verrà norme, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio, in questa direzione. E state certi che noi vi incalzeremo, perché queste sono le misure che servirebbero davvero allo sviluppo, e che le imprese attendono e sollecitano da troppo tempo. Lo approverete questo provvedimento, ma ormai il rituale è frusto, e prima o poi la corda, già sfilacciata, si spezzerà. E questa, almeno, sarà una buona notizia per l'Italia.

*(IdV)*. Signor Presidente, come sempre cercherò di stare nei tempi. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, svolgerà una riunione della Banca centrale europea a Francoforte, la BCE. Nella stessa ci sarà un aumento dei tassi di interesse di riferimento, che passeranno dall'1,25 all'1,50 per cento. Ciò significa che il denaro costerà più caro e che quel rilancio dell'economia difficilmente si potrà realizzare per una parte consistente del Paese, ossia quella parte che coincide con le famiglie, con i mutuatari e con coloro che hanno bisogno di prestiti dalle banche. Proprio ieri, l'ISTAT ha certificato una stagnazione dei consumi (questi sono i dati), poiché la lieve crescita della spesa mensile di uno striminzito 0,50 è stata erosa dall'inflazione, con le famiglie che continuano a tirare la cinghia e a praticare il triplo salto mortale per arrivare, non più a fine mese, ma neanche alla seconda settimana. La spesa media mensile delle famiglie è di 2.453 euro, ma metà dei nuclei familiari sono andati appena sopra i 2.000 euro, con un divario di 1.200-1.300 euro tra il Nord e il Sud del Paese. Un'Italia a doppia velocità, che stringe ancora di più la cinghia rispetto a quelle famiglie che non sono state colpite dalla crisi a quei soggetti che dalla data di entrata in vigore dell'euro hanno sottratto - sono dati questi dalle tasche delle famiglie qualcosa come 187,8 miliardi di euro. Coloro che hanno la possibilità di determinare prezzi e tariffe si arricchiscono sulle spalle della povera gente, assecondati da un Governo strabico, che non guarda all'interesse generale del Paese ma prende semplicemente ordini: e non lo diciamo solo noi, lo ha scritto anche il giornalista Nicola Borzi, non sulla

con costi dei conti correnti pari a 295,66 euro in Italia, rispetto a una media europea di 114 euro. Bisogna

le famiglie? Oppure sono altri e inconfessabili interessi, che coincidono - guarda caso - con i signori del credito,

il secondo atto di norme scritte sotto diretta dettatura dei banchieri è lo smantellamento della legge n. 1996, che regolamentava i tassi di interesse oltre i quali un prestito diventa usurario, per tipologia di prestito. Lo ricordo bene. 1995, l'articolo 644 del codice penale prevedeva lo stato di bisogno per per valutare se vi fosse stato o meno il reato di usura. Era una prova diabolica per il magistrato, perché lo stato di bisogno è difficile da dimostrare. La legge francese prevedeva invece i tassi soglia, una griglia di tassi per tipologia di prestiti (mutui, prestiti personali, *leasing,* eccetera). Vi fu una grande battaglia della società civile. Qualcuno di voi lo ricorda. La battaglia della Confesercenti, il treno contro l'usura che partì dalla Sicilia e arrivò in Piemonte, la Chiesa, il compianto monsignor Di Liegro, padre Rastrelli, le associazioni dei consumatori. La legge n. 108 del 1996 fu approvata, ed è stata una normativa di civiltà giuridica, perché prevede che un tasso, per diventare usurario, debba essere aumentato, rispetto ai tassi medi registrati dal Ministero dell'economia e dalla Banca d'Italia nel trimestre precedente, di uno 0,50 per decreto milleproroghe abbiamo dovuto segnalare, con rammarico, l'obbedienza del Ministero dell'economia agli interessi dell'ABI, l'anatocismo, gli interessi sugli interessi, che sono stati praticati per oltre mezzo secolo dal sistema bancario. Ci sono state sentenze di Cassazione, addirittura due pronunce della Corte costituzionale rispetto a Governi

Nel milleproroghe, invece, la precedente sentenza a sezioni unite è stata cancellata, e si dovrà pronunciare a breve, per l'ennesima volta, la Corte costituzionale, che noi confidiamo

il calcolo del limite oltre il quale si configurava un tasso usurario era fissato da quel meccanismo che ho ricordato. Invece, con questa norma, che è già stata praticata, il Governo aumenta i tassi, aumenta i tassi, fa politica monetaria; i mutui vengono aumentati del 79,8

o vanno a casa o vanno in galera. Sono tutti ancora a piede libero e sono tutti protetti da questo Governo. In conclusione, signor Presidente, mi permetterà il relatore di minoranza,

Mi permetto di non essere d'accordo con lei, perché non si nazionalizza la cricca: questo Governo del fare, trasformato nel Governo del malaffare, legalizza la cricca! Per questo siamo contro, e penso che la maggioranza del Paese spazzerà via un Governo che non rappresenta più

agli atti. Questo decreto-legge, che noi attendevamo con misure per lo sviluppo, non è in grado di dare una risposta adeguata ed imprimere una svolta al *trend* di crescita di politica economica interna del Paese. Ci troviamo in una condizione molto diversa da tutti gli altri Paesi europei e forse anche dagli altri Paesi del mondo. Dal punto di vista della giustizia, tre sono le misure di interesse che il decreto-legge al nostro esame dovrebbe contenere. riguardante la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa e la piena legalità della stessa al fine di favorire il contrasto alla collusione e alla corruzione, la riduzione dei costi assicurando la riduzione del contenzioso, con conseguente maggior efficienza della giustizia e garanzia della concorrenza, prevenendo quindi altresì infiltrazioni mafiose o comunque della criminalità; la seconda, relativa al contrasto alla corruzione e all'evasione fiscale, con conseguente riduzione dei costi per i cittadini e lo Stato e garanzia della concorrenza, all'efficienza e alla rapidità della giustizia civile e penale, per il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese, della competitività, attraverso la concorrenza di mercato e l'attrazione di investimenti, chiudendo contemporaneamente spazi di espansione alla criminalità organizzata. Se così è, *in primis,* si impone - come ha già sottolineato il senatore Agostini - una profonda revisione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in materia di appalti, che ampliano in misura eccessiva e allarmante la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche e delle stazioni appaltanti, rischiando di restringere notevolmente la trasparenza nelle procedure di affidamento di contratti e lavori pubblici senza procedura di gara è aumentata fino a un milione di euro) e il livello di concorrenza tra le imprese operanti nel settore. Come ha giustamente sottolineato il senatore Agostini, se tale misura non sarà corretta, cento degli appalti rischia di essere affidato senza procedura di evidenza pubblica. Contemporaneamente, il decreto-legge prevede un ridimensionato del divieto di ricorrere a subappalti, una previsione che si pone in contrasto con le direttive europee e rischia di esporre l'Italia a procedure di infrazione, oltre ad essere presumibilmente causa di contenziosi giudiziari, con ricadute sulla tenuta, già difficile, del sistema giustizia e, purtroppo, con incremento dei fatti di corruzione. Il decreto-legge che stiamo esaminando perde, inoltre, l'occasione per alcuni interventi indispensabili che proverò a individuare e a elencare. Innanzitutto, il divieto di ricorso all'arbitrato per i contratti pubblici. L'arbitrato ha assunto una valenza tale da essere spesso considerato un momento, seppure ulteriore, dell'esecuzione del contratto e, pertanto, tenuto presente al momento della presentazione dell'offerta

costante delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che porti, con una regolarità quasi assoluta, alla declaratoria di soccombenza della pubblica amministrazione (almeno nel 90 per cento dei casi) rappresenta un dato preoccupante, non solo sotto l'aspetto del detrimento del patrimonio pubblico - dato particolarmente rilevante, in un momento di crisi economica - ma, altresì, di quello del *deficit* di efficienza dell'azione amministrativa che ne costituisce la causa, II costo del giudizio arbitrale è più elevato di quello del giudizio ordinario. Tra l'altro, si potrebbe senza ostacoli alla sola via giurisdizionale prevedendo procedure più veloci presso i TAR e il Consiglio di Stato, anche attraverso l'istituzione di sezioni giudicanti specializzate,

prevedendo, soltanto in tal caso, che questi abbiano requisiti di affidabilità e che siano adottate le modalità più appropriate. A questo proposito, è opportuno richiamare da subito una norma di contenimento di costi e di sana Il divieto di affidamento di incarichi arbitrali, nonché di altri ruoli, ai magistrati, con conseguente riduzione di costi e intervento a favore della trasparenza e della concorrenza. Per quanto riguarda gli incarichi arbitrali, non mi riferisco ai magistrati ordinari, ai quali, per legge, fin dal 1999 è stata vietata la partecipazione agli arbitrati, ma piuttosto ai giudici amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato. Tutto questo crea una commistione non più accettabile, che finisce per creare dei conflitti d'interesse anche istituzionali. A tal proposito, vorrei ricordare che i magistrati amministrativi continuano a svolgere la loro attività istituzionale pur svolgendo l'attività di arbitri, il che significa che «giocano» su due tavoli e, con tutta la correttezza che in linea di massima si vuole riconoscere, non è possibile pensare che in questo caso non si determinino conflitti d'interesse e un ulteriore aumento di costi.

assicurare che i documenti riguardanti la certificazione antimafia non siano semplicemente di autocertificazione, e che ciò valga anche per la posizione contributiva;

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la conversione in legge del decreto-legge in esame vedrà consumarsi, come da noi ampiamente previsto, l'ennesima liturgia del voto di fiducia, su un provvedimento che, carico di attese, a poco a poco si è rivelato per quello che è: una tragica farsa a danno degli italiani, un danno e una beffa alle imprese oneste, che attendevano, con malcelata speranza, tale provvedimento per il rilancio dell'economia del Paese e guardavano a questo momento come ad una possibile occasione di sviluppo. Tale logica sembrava, per certi versi, perfino obbligata per il Governo, se avesse voluto tentare di recuperare un minimo di credibilità con il Paese e agli occhi della comunità internazionale. norme e provvedimenti si poteva e si doveva cercare di uscire da una crisi economica particolarmente dura e non ancora superata nel nostro Paese e su cui il Governo invece colpevolmente si attarda. La risposta al problema della crescita economica ha tradito, quindi, totalmente le attese. Il Governo ormai concepisce il proprio operato finalizzato esclusivamente alla salvaguarda dei propri interessi di bottega, di azienda, come abbiamo visto appena ieri con la norma Mondadori salva-Fininvest prevista nella prossima manovra di finanza pubblica, il cui preventivo disvelamento ha poi costretto al suo ritiro. In questo decreto, denominato impropriamente nella comune accezione «decreto sviluppo», di azioni per lo sviluppo ve ne sono davvero poche. Ancora meno sono le risorse messe effettivamente a disposizione e assai discutibili sono inoltre le norme previste per realizzarle, nella forma, nel metodo, nella qualità e ovviamente nei contenuti.

un intervento che avverto però avere il solo valore della mera testimonianza, dato il livello di attenzione in generale registrato sul provvedimento, cui oggi non sfugge neppure l'Assemblea.

L'articolo 4, con i suoi 19 commi, interviene su ben 32 articoli del codice appalti, che costituisce nei fatti il quarto decreto aggiuntivo al codice, con l'aggravante che contrariamente ai precedenti, possibili perché previsti ed esercitati nei tempi di delega al Governo, il Governo si sottrae totalmente al vaglio parlamentare.

sarebbero potute introdurre modifiche essenziali per rendere quelle norme almeno accettabili. Con il testo in questione si introducono invece degenerazioni a mio modo di vedere insanabili e irreversibili, a partire dal fatto che con queste modifiche al codice - com'è stato ricordato - si sottrae alla trasparenza e alla conoscenza, perfino dell'Autorità di vigilanza, oltre il 96 per cento degli appalti pubblici, innalzando inopinatamente la soglia entro la quale affidare gli appalti a procedura negoziata (la vecchia trattativa privata). Scorciatoie che, come sappiamo bene, sono state spesso fonte di corruzione e clientela, in una parola: occasione di rapporti impropri tra politica e affari. Sono norme che hanno preoccupato e preoccupano per prime le imprese stesse, quelle sane s'intende, quelle gelose della propria autonomia, certe della propria competenza, e che hanno solo da perdere nell'incontro con la politica. Con l'articolo 4 viene poi introdotto il cosiddetto *project* di terza generazione o, a seconda dei punti di vista, di prima degenerazione, in cui si alterano totalmente le dinamiche dei rapporti e delle funzioni tra il soggetto pubblico, titolare della programmazione territoriale, e il soggetto privato, abilitato a presentare la proposta realizzativa dell'intervento. Quello che si consente è un ribaltamento dei piani nel rapporto asimmetrico tra soggetto economico privato e istituzione pubblica, in cui la funzione della programmazione viene di conseguenza alla proposta realizzativa del privato. È facile immaginare che cosa accadrà in ragione di una situazione di enti locali e Regioni strangolati dai tagli ai trasferimenti di questi e dei prossimi anni e che già da tempo si sono visti costretti a reperire risorse *una tantum*, a partire soprattutto dagli oneri di urbanizzazione (leggi consumo ingente di suolo), anche solo per mantenere in essere i propri servizi, a partire dalle essenziali reti di protezione sociale che ben conoscono i cittadini. Infine, giusto per limitarci agli esempi più vistosi e bizzarri di questo provvedimento, si è assistito, con questo articolo, all'introduzione della cultura dei tagli lineari, anche nelle norme sugli appalti, come strumento di contenimento della spesa, come se l'introduzione di un tetto di spesa alle risorse destinabili alle riserve d'appalto o alle varianti in corso d'opera fosse di per sé sufficiente a ridurre o abbattere la lievitazione dei costi che gli appalti pubblici hanno conosciuto in questi anni e non fosse piuttosto un problema di qualità progettuale e di semplificazione del quadro normativo. Viene da pensare che aver confezionato queste norme, nella situazione attuale, significa essere in malafede o essere assolutamente incompetenti, dato che il risultato più probabile che produrranno sarà invece un aumento del contenzioso, proprio quello che con la norma di contrasto alle liti temerarie doveva essere perseguito. Anche per questo provvedimento la sostanza quindi è la solita mistificazione degli annunci a cui ci avete abituato in questi anni. Dichiarate un principio in sé condivisibile, salvo poi negarne i presupposti e perseguire finalità opposte con il provvedimento normativo. In tutto ciò non c'è improvvisazione ma sistematico e scientifico dolo. Il tempo per i risultati attesi che vi eravate impegnati a produrre a partire dalla realizzazione delle opere pubbliche è passato inutilmente e i risultati largamente insoddisfacenti sono sotto gli occhi di tutti. La vostra crisi politica e culturale è manifesta, come la vostra incapacità o impossibilità a realizzare provvedimenti utili alla crescita e allo sviluppo del Paese. Questo provvedimento, colleghi, è anche l'ulteriore sintomo della vostra irreversibile crisi, che finalmente adesso incomincia ad essere percepita e compresa dagli italiani e perfino dai vostri stessi elettori.

intervengo per rappresentare a quest'Aula, così come fatto in precedenza in Commissione, la ferma contrarietà dell'Italia dei Valori nei confronti del cosiddetto decreto-legge sviluppo, ma che - al netto di alcuni risibili interventi, che peraltro noi di Italia dei Valori chiedevamo da tempo - svilupperà ben poco, anzi nulla. Inoltre, colleghi, riteniamo davvero poco corretto nei confronti

testo, ben più importante, costringerà gli italiani, per l'ennesima volta, al sacrificio (sempre sacrifici da richiedere agli italiani). In questo mio breve intervento, colleghi, vorrei soffermarmi sugli aspetti di competenza della nostra Commissione, la Commissione la Commissione istruzione pubblica, beni culturali. All'interno di questo decreto sviluppo, all'articolo 9 del testo, si interviene su alcune questioni importanti quali, ad esempio, al comma 1, i cosiddetti contratti di programma per la ricerca strategica. Anche in questo caso tali contratti, che dovrebbero servire ad aiutare le aree sottosviluppate del Mezzogiorno, mancano di trasparenza e di chiarezza: non si sa in che maniera si vogliono raggiungere determinati obiettivi e come verranno utilizzate le risorse. È abbastanza evidente - ma ormai siamo abituati a questo - che all'interno di questa disposizione normativa ancora una volta il Ministro dell'università sia di fatto commissariato, anche se questa volta non più dal Ministro dell'economia come siamo stati abituati a vedere negli ultimi tre anni e fino ad oggi - ma dal Ministro dello sviluppo economico il quale detterà le condizioni in funzione delle risorse. Continuando, sempre all'articolo 9, con i commi che vanno dal 3 al 16, si introduce il Fondo per il merito che, come quasi tutti sappiamo bene, nasce dalla riforma dell'università, in base alla legge n. 240 del 2010. Attraverso il Fondo per il merito si sarebbero dovuti erogare dal Ministero dal Ministero dell'università i cosiddetti premi di studio, i buoni di studio e i prestiti d'onore agli studenti. Invece, ci ritroviamo di fronte ad un fondazione, partecipata anche dai privati, per fare quello che avrebbe potuto fare direttamente il Ministero dell'università. Nei fatti si istituisce un ulteriore ente, che noi definiamo carrozzone, il quale, tra le altre cose, non avrà neppure le risorse necessarie, considerato che il finanziamento per il solo primo anno è di 10 milioni di euro e di un solo milione per gli anni seguenti. Se non volete ascoltare questo ennesimo appello, dell'Italia dei Valori, date quanto meno retta agli Uffici del Senato

Il tutto per non mettere sotto controllo la vostra maggioranza, una maggioranza ormai a pezzi. In ogni caso, vogliamo ricordare che i tagli al settore dell'università *pre* e *post* riforma ammontano ad oltre un miliardo di euro. Il Governo e le norme approvate dalla maggioranza di centrodestra hanno determinato una condizione per i ricercatori e per la ricerca che chiaramente è di grande difficoltà ed è sotto gli occhi di tutti. È evidente che non si possono fare riforme senza investire risorse economiche e senza dare una destinazione di sviluppo a quelle risorse. Il Governo non lo ha fatto in passato e non lo farà neppure adesso. Per quanto attiene alle disposizioni contenute nei commi da 17 e seguenti, cosa dire? Sono state annunciate come la risoluzione di tutti i problemi del mondo del precariato ma, come sempre accade, non è così neppure questa volta. Prima si è sventrato letteralmente il settore dell'istruzione, con una serie infinite di norme coordinate sempre dal Ministero dell'economia; avete prima tagliato miliardi e miliardi di euro al comparto, lasciando a casa professionisti e precari che fino a quel momento avevano retto il sistema scuola, il sistema università, il sistema ricerca. Poi, quando vi siete accorti

Per non parlare delle sentenze della magistratura, quelle di Genova, sugli indennizzi per la mancata stabilizzazione degli insegnanti. Ancora una volta, accorgendosi che le graduatorie vanno compilate includendo tutti e non escludendo molti, che vanno compilate riconoscendo il merito e non la provenienza geografica, disponete questo piano di assunzioni che non rappresenta altro che l'ennesima riduzione del piano di assunzioni previsto dal precedente Governo, quello del centrosinistra. Avete preannunziato un piano triennale di assunzioni di precari senza investire un centesimo, perché quelle persone che assumerete andranno ad occupare posti vacanti e, dunque, di personale che andrà in pensione. Guarda caso, nel provvedimento non avete indicato neppure i numeri di questo piano triennale di assunzioni. Non potete continuare così. Non potete farlo, perché indicare i i numeri del piano triennale di assunzione significherebbe sapere quanto di più e come spendere. Ma siccome non lo si sa ancora, perché il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti non è in grado oggi di dirvi quanto si può spendere, lasciate la casella in bianco; tanto poi la riempirà l'ennesima manovra di tagli che vi accingete a varare. Per non parlare della deprecabile disposizione contenuta al comma 18 dell'articolo 9, che sottrae il comparto scuola dall'applicazione della normativa europea a tutela dei lavoratori precari e che prevede l'obbligatorietà della trasformazione del del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dopo 3 anni, e che riguarderebbe più di 65.000 precari della scuola. Il Governo che ha presentato questa norma, la maggioranza che l'ha approvata alla Camera e la maggioranza che la approverà qui, vogliono tutti eludere in tal modo le ormai numerose sentenze emesse da diversi tribunali italiani, che nel corso degli ultimi anni hanno riconosciuto ai precari ricorrenti i danni derivanti da una interruzione illegittima dei loro contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, i problemi della scuola non credo possano trovare risoluzione con l'articolo 9 e con questo provvedimento. La verità vera, signor Presidente, è che questa maggioranza e l'attuale Governo considerano le politiche culturali, le politiche legate al mondo della scuola, dell'università e della ricerca come marginali e secondarie rispetto alle politiche economiche e di bilancio. Avete lasciato a casa migliaia di lavoratori precari del mondo della scuola, dell'università e della ricerca, che per noi dell'Italia dei Valori costituiscono un grande patrimonio di cui il Paese non può certamente fare a meno. Avete reso precaria la scuola, avete reso precaria l'università e state rendendo precaria anche la ricerca. Assumetevi la responsabilità di questo sfascio davanti al Paese. Noi continueremo costantemente a difendere quel patrimonio per noi indispensabile, fatto di tante professionalità che si sono adoperate per avere un Paese evoluto e colto, e non un Paese rozzo e abbandonato a questa maggioranza.

Presidente, intervengo intanto per denunciare formalmente in quest'Aula un metodo inaccettabile delle decisioni politiche e delle decisioni di politica economica.

di correzione dei conti pubblici, necessaria per rispondere agli impegni presi con l'Unione europea. Io sottolineo, necessaria per gli impegni presi con i cittadini italiani: non è l'Europa che ci impone l'azzeramento del *deficit*, ma il senso di responsabilità che ci obbliga a mettere i conti a posto. questa manovra, decisa in Consiglio dei ministri lo scorso giovedì, ad oggi, per quello che mi risulta, non è ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Francamente, correttezza istituzionale vorrebbe che il Parlamento, ma anche l'opinione pubblica, potessero discutere, confrontarsi anche in modo serrato, ma su un testo che esiste formalmente. Oggi, a distanza di una settimana, quella

Non sappiamo se e quando il Presidente della Repubblica sarà messo in condizioni di firmare un decreto-legge, e in questi giorni il solito polverone di polemiche che ha all'origine le indiscrezioni, i pezzi di carta, gli annunci e le prese di posizione pro o contro le varie ipotesi che dovrebbero essere contenute nella manovra. Signor Presidente, questo metodo non è accettabile in una normale democrazia, in un regolare rapporto tra Governo, che deve assumere le decisioni, e Parlamento, che deve sostenere o criticare quelle decisioni.

sottobanco e tra le beghe, come capita a ciascuno di noi - una versione della bozza della manovra che sembrerebbe essere quella entrata in Consiglio dei Ministri giovedì scorso. Nella copia che ho,

è tale quand'è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mi riservo di fare commenti più meditati una volta che avrò avuto l'opportunità di leggere il testo vero della manovra.

un'operazione di metodo condivisibile: anticipare le scelte e proiettare l'orizzonte a tre anni, e dunque non nell'immediato. Da quel momento, la manovra avrebbe dovuto mettere i conti a posto per almeno tre anni:

sei manovre perché ogni anno abbiamo fatto il decreto prima dell'estate, che è diventato legge di stabilità in dicembre;

abbiamo sentito dire che il grande rilancio allo sviluppo economico italiano e alla crescita non poteva che provenire dalla modifica dell'articolo 41 della Costituzione.

Poche ore fa, ci è stato detto formalmente dal Ministro dell'economia, in un'intervista, che la manovra

Agisce sul 15 per cento in più di costo della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti? Francamente, c'è da essere molto preoccupati. Sul piano dei numeri,

che, dal 2008 ad oggi, è pari a 118 miliardi di euro: noi avremmo agito sui conti pubblici per una somma di 118 miliardi di euro attraverso le sei manovre cui faccio riferimento. Dopo aver fatto questo, nel DEF di aprile si sostiene che ne occorrono altri 46, da qui al 2014. Quindi, all'incirca nell'arco temporale di una legislatura, avremmo aggiustato i conti pubblici per quasi 160 miliardi di euro, come sommatoria aritmetica della stima dell'effetto della consistenza delle manovre dichiarata dal Governo e riportata dai *media*.

sono finti perché sono misurati sui valori tendenziali degli anni futuri e nascondono in realtà la mistificazione per cui si propongono tagli di spesa lineari, per soggetti, e si tolgono le risorse alle Regioni, alle Province ai Comuni, ai Ministeri, ma riferendosi ai valori tendenziali futuri. Ciò nasconde la realtà, ossia che, rispetto a quanto abbiamo speso l'anno scorso dopo quei tagli lineari, abbiamo aumentato la spesa pubblica, mentre l'aumento delle tasse è vero nel senso che nel DEF di aprile c'è scritto che da qui al 2014 le tasse e le entrate pubbliche aumenteranno di 93 miliardi. Di tale maggiore aumento di entrate, normalmente, in tutte queste manovre, un terzo è destinato a contenere il deficit, due terzi sono destinati a coprire maggiori spese, all'interno delle quali aumentano le spese correnti e vengono tagliati in valore assoluto gli investimenti infrastrutturali. È evidente il risultato masochistico: una rincorsa sul deficit che finanzia aumenti di spesa tagliando gli investimenti non può che deprimere l'economia, creando i presupposti per trovarci tutti insieme, fra un anno o dopo un anno, rispetto ai tre anni passati, di nuovo di fronte alla necessità di tagliare ancora il deficit. L'anno scorso in quest'Aula mi ero permesso di far presente che, dopo la manovra di aggiustamento, quest'anno sarebbero mancati ancora 10 miliardi di euro e - ohibò! - questa mattina la notizia è che l'aggiustamento complessivo della manovra in arrivo sarà di circa 50 miliardi, di cui, guarda caso, 7 miliardi per aggiustare i conti 2011-2012 e gli altri 43 miliardi per il 2013 e 2014. questo trucco che attraversa la storia della Repubblica italiana degli ultimi trent'anni, cioè far finta di tagliare la spesa sui valori tendenziali, scatenare proteste da macelleria sociale e poi ritrovarci, in realtà, con aumenti di spesa non mirati, non decisi dalla politica ma dalla stratificazione genetica delle situazioni pregresse.

mancante. Quando la politica in generale, il Governo il Parlamento, intende sostenere la crescita deve dare il primo esempio,

tutte le medie e piccole imprese italiane debbono essere pagate dalle pubbliche amministrazioni per circa 60 miliardi di euro, la prima manovra a sostegno delle imprese e della crescita è pagare. Certo, c'è un problema di come formalmente incorporare questi debiti nel debito pubblico, altrimenti l'Eurostat ce lo classifica; ma, signor Presidente, chiariamo le cose: innanzi tutto le pubbliche amministrazioni accettino le fatture. è l'unico Paese al mondo in cui le pubbliche amministrazioni non certificano le proprie fatture.

ma sarebbe una linfa finanziaria per le piccole e medie imprese, e successivamente si potrà valutare se un intervento con la Cassa depositi e prestiti possa eventualmente agevolare, accelerare tali pagamenti. riguarda i costi della politica. Signor Presidente, anche qui, giù la maschera: i costi della politica non sono gli stipendi dei parlamentari o i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ma quelle voci di spesa, indicate anche dalla Corte dei conti, e dal governatore Draghi, dove si annidano le truffe, gli sprechi e le malversazioni: quelle decine di miliardi, che in inglese si direbbero *spending* *review* io, usando l'italiano, chiamo fondi perduti, per 40 miliardi di euro all'anno, e acquisti di beni e servizi di tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli appalti, per 150 miliardi di euro all'anno, e oltre!

"succhia" dalle tasche dei cittadini (perché si può succhiare con le tasse, con i*ticket* e taglieggiando i pensionati, cui va garantito il potere di acquisto: riforma Dini del 1995, altro che eliminare o tagliare l'indicizzazione!) Basterebbero 30-40 miliardi di quelle cosacce che ho indicato un minuto fa

di contrastarla e sorreggere l'economia, ma temo di dover dire che gli effetti sono oggettivamente laschi. Ogni manovra è stata anticipata da dichiarazioni dei proponenti - neanche in questo caso credo amplificate dai giornali

Nel nostro Paese la grande crisi non è stata il risultato di un sussulto congiunturale, ma ha creato un nodo storico, che deve essere affrontato con metodi ovviamente più energici rispetto a quelli che altri Paesi europei stanno ponendo in essere. i numeri, più che il commento degli stessi, servano lapidariamente a dire qual è la situazione del nostro Paese e a supportare le ragioni per cui sostengo con vigore e convinzione

perché il segnale forte crea convincimento e fiducia, oltre che le condizioni per cui si ingenerano aspettative positive per l'economia, per le imprese

soggetti che nel nostro Paese reggono sulle proprie spalle il peso della crisi e le aspettative future per la nostra economia.

Siamo stati con gli artigiani un mese fa, e nella mia Regione sono stata con i costruttori ancora lunedì scorso, e viene ripetuto da tutti con molta convinzione. cominciate ad intraprendere le iniziative che non costano, perché da lì avremo il segnale che siete interessati realmente a che le cose vadano meglio.

Quando all'articolo 6 («Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici»), leggo che l'avvio di alcune procedure minimali di semplificazione viene effettuato con decreto del Presente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,

operatori ci chiedono di semplificare gli adempimenti burocratici. Gli artigiani ci hanno detto - era presente il Ministro dell'economia - che sono ben 39 gli accessi che vengono fatti nelle loro aziende, e che quindi il peso

La problematica dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione viene segnalata come una delle patologie italiane radicate nel tempo. Tra le prime iniziative che presi arrivando in Senato, convinta

proponendo confronti su questo molto aperti, la soluzione del problema. Siamo arrivati ad oggi, dopo un'ampia discussione, ad avere un ordine del giorno. Ebbene, io credo che su questa materia non servano né contentini né buffetti. Mi accontenterei - e credo che molti colleghi lo farebbero - di vedere un atto di volontà reale, di mettersi cioè intorno ad un tavolo con i tecnici che nei Ministeri conoscono la materia, che è molto complessa perché ha genesi diverse e quindi richiede soluzioni articolate. Sono tre anni che aspetto che sia proposto, a costo zero, un tavolo con gli interessati per affrontare il problema e che venga proposta una soluzione a tale questione: non un contentino, perché credo che di contentini si muoia, andando avanti di questo passo.

che richiedono un'attenzione e una spiegazione. Vengono aggiunti degli organismi mentre con la mano destra se ne tagliano degli altri. Guardiamo al microcredito. Invito tutti i colleghi ad andare a leggere cos'è l'Ente nazionale per il microcredito.

Non credo che il Paese stesse aspettando con ansia la creazione di un ente, che avrà le risorse adeguate per pagare il personale e gli organi dell'ente. Stessa cosa potrei dire della Fondazione per il merito. Non capisco perché il merito nella scuola, questione che deve essere strutturale, debba essere affidata non alla sorveglianza e alla gestione diretta del Ministero, ma ad un soggetto terzo, di cui per certo sappiamo essere sottodotato rispetto alle finalità,

per noi è uno snodo storico e non un sussulto congiunturale. Si tratta, colleghi, signori del Governo, non di riempire un bicchiere che si è svuotato, ma di sostituire il bicchiere che si è rotto.

ho avuto il privilegio e l'opportunità di poter ascoltare essenzialmente colleghi dell'opposizione che, come sempre accade in queste circostanze, sono protagonisti del dibattito e si esercitano ampiamente in una scarnificazione critica di ciascuno dei passaggi del provvedimento, articolo per articolo, direi quasi comma per comma. Ma, proprio perché ho l'onore di essere uno dei pochi colleghi della maggioranza ad intervenire, mi limito ad alcune brevi riflessioni, riflessioni, ad alta voce, di carattere politico - banalissime, ma temo non superflue - che partono dalla constatazione

Basterebbe ricordare l'intervento, come sempre ricco di contenuto, del presidente Baldassarri, che per otto decimi ha parlato sostanzialmente dell'attesa sostanzialmente dell'attesa manovra, e ben poco di questo provvedimento. Altri senatori hanno fatto lo stesso, anche la gentile collega che mi ha preceduto. Tutto questo non è un caso, è normale.

si inscrive come una componente di una strategia complessiva, che a torto i colleghi dell'opposizione hanno voluto definire inesistente; finché la criticate va bene, ma definirla inesistente, irrintracciabile

delle famiglie, dei cittadini, degli operatori economici e dei risparmiatori una strada, un indirizzo, uno spunto, un'idea alternativa e qualificante, e qualificante, mi pare una pretesa infondata. Infatti, per quanto privo di pregiudizi io abbia voluto ascoltare, se volessi tirar fuori due o tre morali dall'insieme della vostra

che affermano che noi vogliamo smantellare le norme sulla sicurezza sul lavoro o che non siamo sensibili a questa tematica; il che non è vero, ma comunque richiede accumulo di ulteriori norme. Oppure ci accusate di non essere sensibili al tema della protezione dell'ambiente contro l'inquinamento, anche da attività produttive, dagli scarichi, dalle emissioni e da tutto quanto riguarda la vita, i prodotti e i sottoprodotti dell'attività delle imprese, e ci chiedete nuove norme

esemplificativa vi siano organismi del Governo, anche responsabili politicamente, preposti ad intervenire in certi settori o esserne garanzia: volete che si costruiscano nuovi enti, nuove *Authorithy,* in nome dell'indipendenza e dell'autonomia. Criticate il *mix* pubblico-privato, che pure si cerca di sperimentare in più settori con questo provvedimento, e ci rimproverate di e ci rimproverate di essere talvolta persino statalisti, di non dare spazio alla partecipazione delle risorse e degli apporti privati, ma poi siete gli stessi che, un momento dopo, dicono che le politiche del Governo vanno nel senso dello smantellamento delle garanzie di tipo pubblicistico volendo consegnare al privato - come alle volte dite e fate dire in giro nel Paese - settori delicatissimi della vita pubblica. Ci sono cose che sono così contraddette dai dati oggettivi che non vi rendono credibili. Avete parlato molto della scuola, della ricerca,

esclusi dalla riduzione dei trasferimenti l'università, la ricerca, la scuola, il 5 per mille, il Fondo unico per lo spettacolo e le risorse per la conservazione dei beni culturali.

di destra, ci dicono che nella manovra non vi è nessun declassamento dei professori, nessun taglio agli organici, né interventi che vadano a penalizzare le disabilità. Nemmeno uno: tiratelo fuori! Ma non ve ne Ed anche tutto il discorso che avete rispolverato sul precariato non è vero, perché in questi anni è stato anzi aumentato di oltre 4.000 posti il numero degli insegnanti di sostegno,

addormentarci in una situazione non lieve, non leggera e non serena senza un'opposizione di stimolo. Vorrei sapere però i famosi richiami che sempre lodiamo del Capo dello Stato e di altre massime cariche dello Stato che ci dicono che occorrono, tutto sommato, provvedimenti condivisi con un certo qual tasso di consenso convergente per affrontare la pesante situazione economica, sotto certi versi anche sociale, del Paese, in cosa devono tradursi? Non in un'opposizione che non fa opposizione, non in un Governo che non ascolta l'opposizione e le realtà critiche della società. No, al contrario!

Ma se nessun sacrificio di quelli che si configurano vi sta bene - mi riferisco, in particolare, a voi colleghi della sinistra - significa che questo spirito di convergenza non c'è. Se non sta bene che si paghino superbolli sui mezzi di grande cilindrata, se non si possono fare sacrifici scaglionati, e molto, molto, negli anni

della limitatezza dei mezzi, ma anche dalla volontà assoluta di non fare macelleria sociale e anzi di mantenere una solidarietà e una coesione sociale quale nessun altro Paese europeo è riuscito a mantenere in questa crisi, crisi, è una tesi che voi potete propagandare, ma non sostenere con argomenti concreti. Ecco perché dico che questo provvedimento, più o meno sufficiente in tanti suoi aspetti, è tuttavia virtuoso nelle intenzioni e negli strumenti che attiva. Se verrà posto, dunque, il voto di fiducia per le ben note ragioni di carattere tecnico, politico, procedurale che non disconoscete, non sarà certo un abuso, né una scorciatoia, e meriterà un consenso nell'interesse della Nazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, siamo chiamati a discutere l'ennesimo provvedimento sullo sviluppo prodotto da questa maggioranza che, ancora una volta, non affronta i temi strutturali della mancata crescita nel nostro Paese. Non si rimuovono i problemi di fondo della nostra economia che comprimono gli investimenti e l'occupazione, l'occupazione, né si agevolano l'innovazione ed il risparmio energetico, non si sostiene il potere d'acquisto delle famiglie, né si garantisce una reale liberalizzazione dei mercati; anzi si rischia, con gli annunci della prossima manovra economica, di generare insicurezza e paura nei ceti più deboli, a cominciare dai pensionati. Mancate misure che non fanno intravedere, soprattutto se messe in relazione con i contenuti della prossima manovra economica, quella frustata all'economia annunciata dal Premier capace di sovvertire la mancata crescita dell'economia e l'innalzamento costante della disoccupazione. Per raccogliere l'invito del collega Benedetti

Legalità, trasparenza e concorrenza. Dovrebbero essere queste le parole d'ordine utili ad illuminare il nostro cammino in materia di opere pubbliche, infrastrutture e rapporti tra pubblica amministrazione e privati, ma purtroppo, ancora una volta, il Governo, con la scusa della semplificazione, del ridurre i tempi e snellire le procedure, rischia di dare un colpo mortale ad un settore (quello degli appalti) già fortemente in crisi nel nostro Paese. Non si procede con una razionalizzazione del settore che dovrebbe partire, come più volte richiesto dall'opposizione, dal sistema delle imprese e dai sindacati, da una riforma organica del codice degli appalti pubblici capace di eliminare le gare al massimo ribasso, che oltre a destrutturare il mercato delle imprese producono opere di bassa qualità o che non si realizzano,

si procede all'innalzamento delle soglie per il ricorso alla trattativa privata portandolo da 500.000 euro ad un milione di euro e di fatto escludendo dalle procedure concorsuali il 96 per cento delle opere pubbliche. Non a caso su questo punto è intervenuto il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture Giuseppe Brienza, che nella relazione annuale 2010 dichiarato: «Il più delle volte le inefficienze e le diseconomicità sono provocate dall'incapacità degli operatori economici a far fronte agli eccessivi ribassi

di integrare comportamenti opportunistici per rientrare nei propri profitti di impresa». Inoltre, la stessa relazione tende a sottolineare come l'eccessivo utilizzo dello strumento della procedura negoziata,

su un totale di circa di 50.000 imprese sono riuscite ad aggiudicarsi i lavori e di queste 1.400 risultano affidatarie del 50 per cento di tutte le trattative private. Siamo evidentemente in presenza di cartelli d'impresa che soffocano il libero mercato. Questa distorsione del mercato produce ribassi che giungono in alcuni casi al 40-50 per cento della cifra iniziale e che - lasciatemelo dire

le sicurezze, il contratto (che spesso non esiste) delle persone vengono messi fortemente in discussione. È il lavoro nero, è il lavoro per immigrati non regolari, è la fine di ogni civiltà del lavoro! proprio negli ultimi mesi abbiamo registrato nuovamente un incremento degli incidenti, nonostante il rallentamento industriale, in larga misura - a nostro avviso - ascrivibile ad una catena troppo estesa dei subappalti,

le mansioni meno qualificate, le donne, i giovani e gli immigrati. Non sono bastati, quindi, i ripetuti scandali cui abbiamo assistito in questi anni; non sono serviti gli insegnamenti che ci sono venuti dall'uso spregiudicato delle emergenze nazionali, dall'opacità di gestione della Protezione civile. Tutto ciò non è bastato, ma anzi si trasforma in sistema generalizzato e nazionale. Una norma così fatta, oltre a non risolvere i problemi che abbiamo di fronte (quali garanzia sui tempi della realizzazione delle opere, certezza dei pagamenti, qualità stessa delle opere), rischia da un lato di rendere ancora più opaca la cosa pubblica e dall'altro di dequalificare e mettere fuori mercato le imprese sane che in questi anni hanno garantito la sicurezza dei lavoratori, le loro pensioni ed i pagamenti verso l'erario.

il risultato è quello che vedremo domani. ci impegniamo, anche in tempi brevi, a concorrere alla riscrittura di una riforma organica del sistema degli appalti, capace di garantire economie di spesa, qualità, certezza dell'opera, dignità del lavoro; una riforma in grado di coniugare legalità, trasparenza e concorrenza. Voglio aggiungere un'unica osservazione rispetto al pacato ma non convincente intervento di chi mi ha preceduto: si possono fare tante cose, ma non illudete i precari,

Non illudeteli, perché ci troviamo di fronte a una pentola che può esplodere e, se esploderà, voi ne sarete i responsabili.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in esame porta un titolo che ancora una volta apre il cuore alla speranza - diciamo così - e che presto dà delusioni, decreto-legge sviluppo, che dovrebbe essere un provvedimento multisettoriale, dovrebbe avere come comune denominatore la promozione dello sviluppo economico del Paese. Ma ancora una volta dobbiamo sottolineare che si tratta di un provvedimento il cui titolo non corrisponde né ai contenuti, né al metodo che ci vorrebbe per arrivare effettivamente ad un provvedimento di sviluppo per il Paese: un metodo reale di confronto parlamentare, che anche questa volta ci viene negato. Questo decreto, secondo gli annunci che sono stati ripetuti fino a questa mattina, a questa mattina, dovrebbe favorire la ripresa del Mezzogiorno, così come avrebbero dovuto fare i precedenti provvedimenti emanati da questo Governo a maggio e a giugno scorso, tutti riconducibili alla categoria *omnibus*, che pure si proponevano competitività, stabilizzazione e predisposizione di misure anticrisi. La verità è che questo Governo ci ripropone periodicamente sempre le stesse soluzioni, che poi alla fine non sono vere soluzioni. Se quei provvedimenti erano legati alla manovra di finanza pubblica, quello oggi in esame dovrebbe proporre misure di sviluppo, ma la realtà dei fatti è che questo Esecutivo continua a proporre soluzioni anticrisi che soluzioni non sono; come al solito, vorrei dire :tanto rumore per nulla. Si genera appunto una grande illusione, ma alla fine non c'è che il fumo di annunci cui non seguiranno vere soluzioni. un decreto sviluppo che dovrebbe affrontare e risolvere i problemi di un Paese che sta rischiando tanto. Le statistiche, i dati che ci forniscono l'ISTAT e la stessa Banca d'Italia che la disoccupazione è pari all'11,8 per cento, senza tener conto dei circa due milioni di individui che non studiano, non lavorano e che quindi non sono calcolabili. La percentuale sale a quasi il 30 per cento in alcune zone del Paese, come il Mezzogiorno. Questi dati ci danno la misura di quanto la situazione sia veramente insostenibile. Il nostro è un Paese che non cresce più, in cui diminuiscono i redditi, i consumi e l'occupazione; un Paese fermo che, più che svilupparsi, sembra decrescere e dove gli unici numeri che sembrano crescere sono quelli della disoccupazione, dei precari, delle tasse da pagare e dell'indebolimento del Mezzogiorno. Entrando nel merito del provvedimento, non passano certo inosservate le disposizioni che dovrebbero contenere misure positive per il Sud e sollevare un po' la situazione del nostro Mezzogiorno. Mi riferisco, in particolare, alle misure contenute nell'articolo 2, specifico al credito d'imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno e al credito d'imposta per gli investimenti al Sud. Certo, detta e letta così, dovrebbe essere una misura molto positiva una misura molto positiva che richiama quella che il Governo Prodi aveva varato a favore dell'occupazione nel Mezzogiorno e che era stata velocemente cancellata all'inizio della legislatura da questo Governo.

aspettare un'autorizzazione alla individuazione delle fonti di copertura da parte della Commissione europea e, come si sa, ci sarebbero voluti uno o due anni.

al Governo di rendere operativa la misura con ricorso immediato ai fondi FAS, anche in attesa di una risposta della Commissione europea. Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per gli investimenti al Sud, la modifica apportata dalla Camera prevede una clausola di salvaguardia che specifica che i crediti saranno concessi nei limiti degli stanziamenti esistenti; quindi, presumibilmente si ricorrerà sempre al FAS. Noi avremmo presentato (uso il condizionale perché, naturalmente, il fatto di privarci della possibilità di utilizzare il confronto parlamentare per migliorare il provvedimento impedirà l'esame emendamenti) un ulteriore rimedio volto a correggere la copertura finanziaria, al fine di rendere tali disposizioni immediatamente attivabili. Si era proposto di utilizzare da subito le risorse liberate dal FAS del ciclo di programmazione 2000-2006, che ammontano complessivamente a circa 11 miliardi di euro:

provocare delusioni immediate al Mezzogiorno: basti pensare a quello che non è stato il piano per il Sud che, anzi, ha avuto come unico effetto quello di puntare sulla riprogrammazione dei fondi europei del quinquennio

di una ulteriore difficoltà alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno che, di fatto, da questa scelta subiranno

come ho già avuto modo di sottolineare durante il dibattito in Commissione, il cosiddetto decreto sviluppo si presenta come un insieme di norme eterogenee - molte delle quali non hanno nemmeno i requisiti di necessità e urgenza - delle quali si può legittimamente dubitare che abbiano una qualche efficacia nel rilancio della crescita e della produttività del nostro sistema Paese. Peraltro, la necessità di predisporre un'ulteriore pesantissima manovra, come quella che ci troveremo a discutere a partire dalla prossima settimana, indica che ben altre sono, o dovrebbero essere, le urgenze da affrontare. Questo decreto è l'ennesimo interventino parziale, frutto di una navigazione a vista, che sembra ormai l'unica che la maggioranza si può concedere: si dipana in 10 articoli, più di 300 commi, senza minimamente procedere sulla strada delle riforme, anzi, in alcuni casi, complicando ancora di più il quadro burocratico, come nel caso della normativa sugli appalti, o prevedendo misure di entità risibile, come i 10 milioni di euro che dovrebbero andare a premiare il merito scolastico, stanti i tagli apportati negli ultimi anni alla pubblica istruzione. Nessuna disposizione poi è volta a sanare il *gap* occupazionale di genere, che spesso diventa semplicemente*gap* sociale, e a rimediare allo scippo dei quattro miliardi derivanti dall'aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego, e che per legge avrebbero dovuto essere destinati esclusivamente al finanziamento delle politiche sociali e per la conciliazione lavoro‑famiglia. Per quanto concerne le disposizioni in materia di lavoro, si deve innanzitutto rilevare un problema già sollevato alla Camera ma solo parzialmente risolto, che presenta tratti persino imbarazzanti. Mi riferisco all'articolo 2, che contiene svariate espressioni scritte in stile colloquiale informale, di cui non è possibile stabilire la portata normativa, il significato e l'utilità. Nel comma 1, per esempio, si fa riferimento a misure la cui scelta è di competenza dell'Unione, che non è quindi nella possibilità del Governo programmare; come pure si utilizza l'espressione «per cominciare», che non vuole dire nulla dal punto di vista legislativo. Al comma 8 è scritto che le risorse per il credito d'imposta spettanti a ciascuna Regione sono distribuite tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari. Ciò farebbe anche intendere che è volontà del Governo punire quelle Regioni che in passato non hanno speso, o ben speso, i fondi strutturali comunitari, attribuendogli risorse in misura inferiore ad altre Regioni. Una tale previsione non avrebbe senso se la *ratio* del provvedimento è quella di favorire l'occupazione e la stabilità. Oltre a ciò, risulta altresì evidente come sia necessario individuare anche una diversa copertura finanziaria, certa e subito disponibile per consentire all'incentivo di funzionare. Infatti, il decreto non ascrive all'articolo 2 effetti sui saldi di finanza pubblica; ciò crea margini di incertezza relativi alle risorse a disposizione dell'incentivo, nonostante la copertura individuata sarebbe potenzialmente superiore ai costi del credito d'imposta. Il finanziamento dell'incentivo alle assunzioni pone dei problemi. Con un gioco di parole si potrebbe dire che se da una parte ci sono i soldi, dall'altra non c'è la copertura; infatti, il comma 6 afferma che il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, cioè fin dal pagamento dell'F24 di giugno 2011, quindi anche da subito ed entro i successivi 3 anni; ma il comma 9 copre il credito con risorse di fondi europei su cui l'Unione europea deve dare un consenso preventivo. Ciò vuol dire che, se il consenso ci sarà, sarà necessario attendere i tempi tecnici e burocratici perché le istituzioni dell'Unione esprimano questo consenso, in contrasto con quel possibile utilizzo immediato del credito che sembra consentito dal comma 6. In caso di parere negativo, inoltre, si verrebbero a creare molti problemi giuridici, perché l'impresa che ha assunto lavoratori a tempo indeterminato avrebbe acquisito un diritto a godere del credito d'imposta, che non potrebbe esserle revocato. Un ulteriore elemento di ostacolo burocratico è dato dal fatto che i limiti del finanziamento di quest'incentivo, Regione per Regione, saranno determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 8, che - per ovvie ragioni - è ipotizzabile non venga adottato prima della pronuncia dell'Unione europea. Anche per questi motivi, evidentemente il comma 9 non contiene una quantificazione delle risorse necessarie e rese disponibili per realizzare questa misura incentivante. Se l'Unione europea approva, potranno essere rese disponibili maggiori risorse; se non approva, queste saranno ridotte, probabilmente annullando la portata del beneficio, perché dovranno provenire dal FAS. Il nuovo credito d'imposta per le assunzioni al Sud, infatti, sfrutta le risorse UE destinate a quei territori dal fondo sociale europeo e dal fondo europeo di sviluppo regionale. Nel caso in cui l'Europa - come dicevo prima - non autorizzasse l'utilizzo di questi fondi per questo credito d'imposta o se essi non fossero sufficienti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a ridurre la dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate, in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica. Infine, non va sottovalutato che, per il principio dell'addizionalità, in corrispondenza alle quote di risorse comunitarie che transitano dai fondi strutturali per il raggiungimento di ciascun obiettivo delle politiche di coesione e sviluppo, si prevede un ammontare pressoché pari di cofinanziamento nazionale, che transita dal fondo di rotazione per l'attuazione di politiche comunitarie. Questo meccanismo, se trovasse applicazione anche nel caso di tale credito d'imposta, sarebbe in grado di paralizzare la misura introdotta, considerati i magri bilanci di Stato e Regioni. Noi, come Gruppo dell'Italia dei Valori, abbiamo presentato vari interventi emendativi, tra i quali proponiamo l'introduzione di una serie di misure a favore delle donne, che mi stanno molto a cuore: incentivi fiscali in favore delle imprese che assumono donne, in particolare nel Mezzogiorno, e la proroga e l'incremento del credito d'imposta per l'occupazione, introdotto con la finanziaria 2008;

finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome; il rifinanziamento del fondo per gli asili nido, di cui sempre alla finanziaria del 2007, al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro quest'anno, in attuazione dell'obiettivo di Lisbona della copertura territoriale del 33 per cento, e incentivi a tutte le aziende che istituiscano al loro interno un asilo nido; misure volte a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di tutte le donne disabili, indipendentemente dalle cause che ne hanno originato la disabilità. Signor Presidente, credo che avrebbero dovuto essere messi in campo provvedimenti come questi, se si fosse voluto sul serio iniziare un cammino di ripresa e sostegno all'Italia provata dalla crisi.

signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ci è voluto il quarantaquattresimo voto di fiducia della Camera per approvare il testo del decreto sviluppo, che giunge oggi alla discussione del Senato. Il testo è stato licenziato dalla Camera dei deputati con 308 voti favorevoli: questi stessi numeri sono il segnale della profonda debolezza del Governo e non della sua forza, come invece il Presidente del Consiglio vorrebbe far credere agli italiani. Il clima politico che imperversa nella maggioranza e le tensioni che la segnano fanno ritenere che il provvedimento *omnibus* di semplificazione e di presunto rilancio economico giunga alla discussione in Senato in modo assolutamente blindato. Persistere in questo atteggiamento sarebbe un errore gravissimo. Tuttavia, se così fosse, dimostrerebbe, se ancora ce ne fosse bisogno, che una maggioranza tenuta insieme solo da un disegno di forzata convenienza politica, è doppiamente dannosa per il Paese: è dannosa perché non riesce a perseguire un qualche progetto coerente sul quale confrontarsi; è dannosa perché questa maggioranza è costretta a governare limitando, bloccando, contenendo ogni discussione ed ogni confronto con l'opposizione, così come con le forze economiche e sociali del Paese. Giorno dopo giorno, le tensioni della maggioranza, le contraddizioni, le diversità culturali, le piccole e grandi guerre di potere, nonché la quotidiana preminenza dei casi giudiziari personali (e non solo) del Presidente del Consiglio sugli interessi generali del Paese sono apparsi via via sempre più chiari a fasce ampie di quell'elettorato italiano che, che, prima con i risultati della consultazione amministrativa e poi - e forse principalmente - con gli esiti referendari, ha segnato un momento di consistente frattura tra Governo e Paese. È in questo clima che nasce il decreto sviluppo e si appresta a prendere forma una manovra finanziaria da quasi 50 miliardi di euro che affonderà pesantemente le mani nelle tasche di tutti gli italiani. Ancora una volta ci troviamo di fronte un documento sostanzialmente disarticolato, come tutta la produzione normativa di questa maggioranza, incapace di esprimere non dico un disegno unitario d'intervento, ma anche semplicemente un quadro organico di priorità. Ritengo che, in un momento finanziariamente così difficile, si sarebbero anche potuti fare interventi utili di semplificazione e di miglioramento della competitività del sistema Italia a costo zero, ma a condizione di saper costruire una rete di interventi organici e in sinergia tra di loro; interventi che avessero chiari alcuni obiettivi: semplificazione, qualità, efficacia, liberalizzazioni, ragionevole sostegno della concorrenzialità. La dizione «senza ulteriori costi per la pubblica amministrazione», da sola, è insufficiente e si traduce ancora in tagli lineari. Occorrerebbe invece saperla declinare con la traslazione di alcune risorse, cioè facendo scelte chiare in termini di priorità. Non mi sembra sia questo il caso del decreto-legge oggi in discussione, costruito con il metodo stantio degli interventi *omnibus*, senza un coerente ed incisivo filo conduttore, qualche volta addirittura in contraddizione. Proprio per questo motivo il Gruppo del Partito Democratico ha ritenuto indispensabile presentare oltre 100 emendamenti (forse ne avrebbe voluti presentare di più), solo per tentare di correggere aspetti contraddittori che finiscono per soffocare la concorrenza o annullano semplificazioni introdotte dando vita a nuovi tortuosi percorsi di gestione. È il caso della modifica di alcune norme sugli appalti dove, tra l'altro, la maggiore discrezionalità rischia di trasformarsi in nuove forme

e necessaria riflessione sul rapporto tra enti pubblici e cittadini, un rapporto che oggi risulta solamente autoritario, iniquo e carissimo per i cittadini e spesso oneroso ed inefficiente per gli stessi enti. La semplificazione, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti sono cose estremamente serie e non possono essere ridotte ad etichette per la propaganda. Il Patto di stabilità va salvaguardato, lo impone la situazione e rappresenta un criterio ragionevole per la tutela degli equilibri finanziari. Ma perché continuare a punire gli enti virtuosi? Perché, con la dovuta attenzione e ragionevolezza, non liberare risorse utili per dar respiro ad alcuni settori della nostra economia? Perché non premiare gli amministratori più accorti? Ancora un altro esempio: la stabilizzazione del 5 per mille. Si tratta di una misura che non solo premierebbe, in base all'autonomo giudizio dei cittadini, l'operato di molte, meritevoli organizzazioni *no profit*, ma agirebbe anche da stabile moltiplicatore delle risorse, considerando che la totalità degli interventi che renderebbe possibili ricadrebbero direttamente nella ricerca o, in particolare, in moltissimi settori della società civile. Per quanto riguarda le attività produttive, e in particolare il turismo, vorrei soffermarmi sull'articolo 3, un testo partito male, fortunatamente modificato alla Camera a seguito di una fortissima opposizione in Parlamento e nel Paese. Sono stati infatti soppressi i commi originari 1, 2, 3 e quelli relativi alle concessioni demaniali marittime che istituivano un diritto di superficie sul demanio prima di 90 anni, poi di 20, poi forse di 15, in un quadro di totale confusione che non risolveva i problemi dei balneari, ma li cacciava in un'incresciosa situazione di discredito da parte di tutte le associazione ambientaliste e dell'intero Paese. Ancora pressappochismo e confusione, eppure si tratta di una quota rilevante dell'economia turistica del nostro Paese. Proprio con questo articolo siamo di fronte ad un esempio della totale disorganicità e superficialità degli interventi dell'attuale Governo. È altrettanto evidente che la proposta dei distretti, fortunatamente corretta alla Camera, di per sé non è sufficiente per affrontare la questione: occorre un'iniziativa di ben altro spessore e di ben altra organicità. È chiaro che si è persa un'altra occasione. Ora, nonostante un quadro politico assai complesso e difficile, siamo impegnati a lavorare per una legge quadro, essenziale per affrontare organicamente tutta la questione, in particolare affinché le attività turistico-ricreative-balneari siano escluse, in analogia con altri tipi di attività, dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein nell'ordinamento italiano. Torno quindi a chiedere, anche in questa occasione in cui

quali fattori di esclusione, del sussistere della libertà di stabilimento in ragione della vastità delle risorse naturali presenti lungo le coste italiane e della conseguente possibilità di rilascio di nuove concessioni. L'articolo 3 è l'unico articolo che riguarda le imprese